vuole tenersi un po' lontano da argomenti indubbiamente molto pesanti e molto delicati, che però segneranno per una lunga fase la vita politica e economica del nostro Paese.

viva del nostro Paese - andranno assunti nel passaggio 2014-2015. Bisogna cominciare a ragionare, e forse anche a formulare delle politiche che nel frattempo, fino al 2014-2015, a prescindere da chi sarà maggioranza e opposizione, vadano nella direzione giusta per quanto riguarda la messa sotto controllo delle grandezze della finanza pubblica, e anche delle scelte di sviluppo.

marzo in sede di Consiglio dell'Unione europea), debba essere presente in quest'Aula il ministro Tremonti, per ragionare con il Senato su alcuni dei dati fondamentali che stamattina sono stati proposti sia dal relatore, senatore Azzollini, che nella relazione di minoranza del collega senatore Morando. Venga innanzitutto il Ministro anche ad assumere alcuni impegni di carattere nazionale per quanto riguarda il documento che è stato sottoscritto dal presidente del Consiglio Berlusconi nei giorni scorsi e che impegna il Governo italiano, e naturalmente in prima persona il suo rappresentante - leggo testualmente dal documento documento - «a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'Unione europea fissate nel patto di stabilità e crescita». E ancora:

quali ci siamo impegnati come Paese attraverso la rappresentanza del ministro Tremonti e del Presidente del Consiglio, si rende conto che a partire dal 2014 l'Italia si impegna in questo contesto ad alcune azioni molto robuste, in primo luogo quella di mettere sotto controllo

metà) deve rientrare nel corso di questo periodo. Ciò significa che, se operiamo sui 900 miliardi, che sono sostanzialmente eccedentari, dobbiamo fare manovre che solo a questo fine impegneranno il bilancio dello Stato ogni anno per importi di 42-43 miliardi Certo, si può aggiungere che è evidente che l'impegno più importante sarà quello relativo ai primissimi anni, poiché il peso sarà maggiore, mentre man mano che ci allungheremo nelle scadenze, sia perché l'inflazione sarà già in azione, e quindi alleggerirà alleggerirà il debitore (in questo caso lo Stato), sia perché ci sarà una riduzione del montante, l'impegno sarà minore. È però evidente che di questo stiamo parlando.

tempo (quindi nell'arco di cinque, sei anni) l'impegno a cui l'Italia già sottosta (e cioè l'aggiustamento dello 0,50 sullo strutturale ogni anno, che è quello a cui siamo sottoposti oggi, dopo il 2005) e l'impegno che ricordavo prima, di una manovra che riguarda il 5 per cento sul debito eccedente, sostanzialmente si equivalgono. Ma stiamo parlando di questioni di grandissimo rilievo e di grande importanza.

giustamente io dico, il ministro Tremonti insiste da molto tempo), e cioè il fatto che gli aggiustamenti dell'Italia debbano essere parametrati rispetto ad alcuni elementi positivi che il nostro Paese possiede a differenza di altri Paesi. Mi riferisco al livello del risparmio privato che, come sappiamo, è altissimo; mi riferisco al fatto al fatto che abbiamo già realizzato la riforma nel settore previdenziale e pensionistico e al fatto che l'Italia ha altri *asset* importanti nel patrimonio pubblico che potrebbero contribuire, con operazioni straordinarie, a ridurre la massa su cui dobbiamo intervenire attraverso le manovre annuali. Tutti elementi di grandissimo rilievo che riguardano la composizione qualitativa, come si dice tecnicamente, del debito pubblico, ma che è bene che vengano affrontati nel merito.

quali strumenti il bilancio pubblico può mettere a disposizione di settori che tutti riteniamo strategici per lo sviluppo del Paese (dal campo della formazione, al campo dell'istruzione

anche l'impatto complessivo macroeconomico sul sistema europeo, non solo italiano, nel caso in cui tutte queste manovre vengano messe in atto contemporaneamente. Ci sono infatti economisti che sostengono che il rischio di una componente recessiva nel caso di manovre fatte tutte in contemporanea può essere di un qualche rilievo. Il secondo punto su cui sarebbe importante avere la valutazione del Ministro riguarda l'articolo 4 del provvedimento in esame: il monitoraggio sull'andamento delle finanze pubbliche da parte del Parlamento

in cui ci rinfacciamo reciprocamente le cose, ci diciamo che le cose non vanno e che le grandezze sono fuori controllo, oppure, potremmo fare una discussione di merito rispettando una sorta di patto tra di noi (perché poi - vivaddio - le alternanze di governo ci sono sempre). Fare una discussione di merito significa disporre di uno strumento tecnico che consenta al Parlamento quell'analisi specifica sull'andamento dei conti pubblici di cui c'è bisogno.

24-25 marzo circa le effettive risultanze di questo dibattito che vede il nostro Paese impegnato

un altro dato. La Francia, uno dei nostri diretti concorrenti, nel triennio 2009-2011 ha peggiorato il deficit di 220 miliardi di euro, più di 70 miliardi di euro l'anno. non è male quello che siamo riusciti a fare, pur in un periodo di estrema difficoltà. Anche il PIL è cresciuto l'anno scorso più del previsto

al 43,3 del 2007. Nel biennio 2005-2007, quando il PIL cresceva, siamo riusciti nell'operazione, non certo buona, di far crescere la pressione fiscale di un punto. Invece, il fatto di essere riusciti in anni negativi

il commissario Olli Rehn ha detto ufficialmente che la vera novità per quanto riguarda il nostro Paese è la considerazione effettiva, all'interno dei parametri di valutazione del debito,

è a conoscenza di chi in 5a Commissione non si occupa solo del bilancio dello Stato. Purtroppo, ormai la componente discrezionale di quegli 820-830 miliardi di uscita

alle Regioni come enti di programmazione e di spesa; pertanto, a nostro avviso, è ancora più rilevante e urgente completare in tempi rapidissimi la riforma del federalismo fiscale, proprio perché abbiamo di fronte una sfida molto importante che ci obbliga a qualificare meglio la spesa

completare la riforma federale, per dare ai governatori delle Regioni la responsabilità di avere entrare sane e giuste con cui finanziare una spesa sana e giusta con il tetto dei costi standard.

alla Camera la proposta è stata approvata all'unanimità ed il relatore era appartenente al nostro partito, non si capisce perché abbiamo questo atteggiamento

molto positivo, va detto che in questi giorni sono subentrate alcune novità; in particolare,

sui quali si devono attestare i Governi dei vari Paesi per affrontare la *governance* europea,

Presidente del Consiglio, così come quella di altri Capi di Stato e di Governo. Si dà il caso che questa posizione e questo documento, molto dettagliato peraltro,

e puntuali. Da questo punto di vista, noi non faremo un passo indietro, se non in un ragionamento che abbiamo avviato, e rispetto al quale ci rendiamo conto del senso di responsabilità e della misura che ci vuole in questo momento.

crescita. Se si potesse andare a quella riunione con un voto unanime, sarebbe un fatto molto positivo. Ma, se si vuole andare a quella riunione con un voto unanime, bisogna che il Governo si assuma la responsabilità di dare un segnale che vada nella direzione di accogliere alcune delle nostre proposte (che abbiamo formulato con emendamenti in maniera molto puntuale e molto precisa) e, al tempo stesso, bisogna

per cercare di costruire a più voci, quindi anche con il nostro contributo, una linea da portare avanti in Europa. Io credo che questa sia una posizione del tutto

a seguito dell'ampio dibattito, sviluppatosi in relazione alla definizione della nuova strategia dell'Unione europea per fronteggiare la crisi finanziaria, le istituzioni europee hanno presentato iniziative volte a rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei Paesi membri. In particolare, l'avvio del cosiddetto semestre europeo, stabilito dall'ECOFIN già a partire dal 2011 impone all'Italia un adeguamento del ciclo e degli strumenti di programmazione finanziaria al fine di consentire un pieno allineamento tra la programmazione nazionale e quella europea. In questa prospettiva si pone la proposta di legge all'esame di questo consesso, sottoscritta da rappresentanti di diversi Gruppi di maggioranza e opposizione, e votata all'unanimità dalla Camera dei deputati

con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea ed in particolare con il "semestre europeo", nell'ambito del quale l'Italia è chiamata a presentare il proprio Programma di stabilità e convergenza e il Programma nazionale di riforma. In tal senso deve leggersi anche la riconferma del principio del concorso di responsabilità di tutte le amministrazioni pubbliche nel perseguimento degli obiettivi economico-finanziari, da realizzarsi secondo principi di armonizzazione e coordinamento con le linee guida delineate dall'Unione. il primo obiettivo che si intende cogliere è quello di anticipare la presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), che sostituisce l'attuale Decisione di finanza pubblica (DFP), al 10 aprile di ogni anno per consentire al Parlamento di approvarlo entro il 30 aprile. Il DEF conterrà gli schemi del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma che devono essere presentati in Europa entro il 30 aprile, documenti di centrale importanza nella logica di rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione. In tali documenti sono contenuti gli obiettivi delle politiche economiche che, nell'impostazione europea, devono rimanere fermi anche al variare dell'entità delle manovre con l'oscillazione delle previsioni. Tutto questo ha anche implicato una rivisitazione delle modalità di coinvolgimento delle autonomie territoriali, nonché una diversa strutturazione della Nota di aggiornamento, da presentare a settembre, confinata - come già detto - alla modifica delle previsioni, fermi rimanendo quindi gli obiettivi fissati ad aprile. Altro passaggio significativo del testo in esame è quello riguardante i limiti della dinamica della spesa e del rafforzamento delle politiche di risanamento. In tal senso vanno viste le misure che impediscono, nella legge di stabilità, di introdurre aumenti di spesa con copertura sul miglioramento del risparmio pubblico; un incremento di spesa corrente, quindi, deve trovare coperture con misure contenute nella stessa legge di stabilità e non può più attingere a risorse dovute al miglior andamento a legislazione vigente. si sposano con l'altra innovazione che prevede che tutte le maggiori entrate, rispetto alle previsioni, debbano andare a beneficio della riduzione del deficit*,* in linea con l'indirizzo comunitario di contenimento della spesa e riduzione del debito. Senza dubbio, quindi, rispondendo alla domanda posta questa mattina dal relatore di minoranza, senatore Morando, il Governo e il Parlamento italiano hanno partecipato e partecipano in maniera attiva al processo di nuova *governance* della finanza pubblica europea. Va ricordato infatti come il Governo italiano sia stato coerente nei vari passaggi critici che l'Unione europea ha dovuto affrontare a seguito della crisi dei mercati finanziari degli anni scorsi e dell'attacco ai debiti sovrani di importanti Paesi membri, circostanze che hanno messo in discussione la stessa prosecuzione del percorso unitario. L'Italia si è collocata tra i Paesi virtuosi,

oggetto in questo momento di importanti discussioni in sede comunitaria sul tema dei parametri e dei vincoli da considerare nella stima e nella comparazione dei livelli di debito. È noto che l'Unione sta considerando positivamente le proposte italiane di inserire nella valutazione del debito di un Paese anche il debito delle famiglie e la solidità del sistema bancario, fattori che sono stati decisivi per la tenuta del nostro sistema economico-finanziario nel corso delle ultime crisi. Questo non vuol dire che poi il nostro Paese non debba prestare sempre attenzione sullo *stock* di debito pubblico. L'Italia è comunque tra i Paesi che hanno modificato più velocemente le proprie normative contabili per tenere conto delle decisioni europee. Anche questo, senza dubbio contribuisce a dare credibilità alla decisione di finanza pubblica italiana.